il disegno di legge oggetto del nostro esame è già stato approvato dalla Camera e riguarda un accordo tra l'Italia e il Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale. Il testo ricalca il modello predisposto dall'OCSE nel quadro delle iniziative per la trasparenza fiscale ed è pienamente in linea con gli orientamenti fatti valere dall'Italia nelle diverse sedi multilaterali per il rafforzamento degli strumenti di contrasto al fenomeno della evasione fiscale internazionale. altre esaminate in questa sede, ha lo scopo di favorire la cooperazione fra le amministrazioni delle due Parti attraverso uno scambio di informazioni che garantisca adeguati livelli di trasparenza. Il Protocollo annesso, inoltre, consente di conseguire effetti equivalenti a quelli previsti dal modello OCSE di convenzioni contro la doppia imposizione Il testo risponde pienamente ai requisiti previsti dalla recente normativa italiana in materia di rientro dei capitali, consentendo ai contribuenti italiani con disponibilità finanziarie a Montecarlo di fruire di una più agevole regolarizzazione. Composto di 14 articoli e da un Protocollo, l'Accordo definisce innanzitutto le imposte oggetto del possibile scambio informativo, cioè per l'Italia, IRPEF, IRES, IRAP, imposta sulle successioni, quella sulle donazioni e le imposte sostitutive. Vengono regolate le modalità di svolgimento dello scambio di informazioni, disciplinando nel dettaglio le tipologie di informazioni che possono essere richieste. Viene anche previsto il superamento del segreto bancario, conformemente agli *standard* dell'OCSE in materia. Gli articoli 6 e 7, che disciplinano le verifiche fiscali nei rispettivi territori, consentono anche di descrivere le ipotesi in cui sia possibile per una delle Parti sottrarsi alla richiesta di informazioni. Importante anche l'articolo 12, che contiene disposizioni per eliminare i casi di doppia imposizione, prevedendo in particolare l'applicazione del credito d'imposta secondo la formulazione *standard* utilizzata in genere dall'Italia e regolamentando i casi di doppia residenza fiscale. Il disegno di legge di ratifica si compone di tre articoli che dispongono l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore. Il testo non comporta spese e non determinerà minori entrate. La Commissione non ha ravvisato alcun profilo di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e, anzi, ritiene che il testo rappresenti un completamento degli obblighi internazionali

verbale, preciso che, avendo dichiarato che avevo sbagliato nel procedere alla votazione, si intendeva annullata anche la verifica del sostegno alla richiesta di votazione elettronica, perché non potevamo procedere al voto.

sviluppato sul modello predisposto dall'OCSE e serve a rafforzare gli strumenti di contrasto al fenomeno dell'evasione fiscale internazionale attraverso uno scambio maggiore di informazioni, teso a garantire livelli di trasparenza. Per questi motivi il

*relatore*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame riguarda la cooperazione in materia di cultura e istruzione tra l'Italia e la Repubblica ceca. Vorrei in primo luogo sottolineare che il testo in esame è d'iniziativa parlamentare anche se riproduce un disegno di legge d'iniziativa governativa che era stato presentato nella scorsa legislatura senza però essere mai discusso. L'intesa sostituisce i precedenti accordi bilaterali ed è finalizzata a fornire un quadro aggiornato di riferimento per le iniziative di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica fra le parti. La necessità di un aggiornamento deriva dalla positiva evoluzione degli scambi culturali e scientifici tra i due Paesi avutasi negli ultimi anni e soprattutto dalla considerevole richiesta di lingua e cultura italiana nel territorio della Repubblica ceca. I dati relativi all'interscambio culturale segnalano infatti un considerevole aumento del numero di accordi interuniversitari tra atenei italiani e controparti ceche, a testimonianza del crescente interesse reciproco a livello accademico. Numerose sono, in tutto il territorio della Repubblica ceca, le attività di promozione della lingua e della cultura Italiana, a partire da quelle promosse dall'Istituto italiano di cultura di Praga e dalla «Dante Alighieri». La lingua italiana viene insegnata anche presso sette università ceche, mentre a livello di insegnamento secondario si segnalano il liceo italo-ceco Ustavni, che ha che ha attiva sin dal 1991 un'apposita sezione bilingue, e alcuni altri istituti, tra cui il liceo linguistico Sazavska, che, tra le varie lingue straniere oggetto dei propri corsi di studio, sta ampliando e diversificando la propria offerta formativa in lingua italiana. L'italiano è inoltre presente anche a livello di insegnamento primario e di scuola secondaria di primo grado e a livello prescolare. L'Accordo consentirà di promuovere ed incentivare iniziative, scambi e collaborazioni in ambito culturale, scientifico e tecnologico mediante l'organizzazione di convegni e l'attribuzione di borse di studio, facilitando altresì la cooperazione nella conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico e archeologico, con particolare riguardo al contrasto dei trasferimenti illeciti di beni culturali ed alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Il testo si compone di un preambolo e di 20 articoli, che individuano le finalità ed i settori della collaborazione, oltre che le modalità di esecuzione della cooperazione. Particolare rilievo assumono le disposizioni relative ai distinti ambiti di collaborazione a partire dalla cooperazione fra istituzioni universitarie, mediante l'avvio di ricerche congiunte e un'offerta reciproca di borse di studio in settori considerati prioritari dalle parti. Vengono anche promosse e facilitate le attività delle istituzioni culturali di un Paese all'interno della realtà culturale dell'altro e favorito lo sviluppo di attività comuni tra i propri istituti e le istituzioni culturali del Paese ospitante. L'articolo 9 esplicita l'impegno delle parti a contrastare il traffico illecito di beni culturali, anche nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione UNESCO in materia. L'Accordo disciplina, inoltre, le forme di cooperazione scientifica fra istituti, centri di ricerca scientifica e università dei due Stati mediante scambi di documentazione scientifica e tecnologica, scambi di esperienze e di visite di docenti, ricercatori e tecnici. Il testo stabilisce anche il reciproco impegno delle parti a proteggere la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i diritti connessi, in particolare all'articolo 14. L'attuazione dell'intesa è rimessa, come per altri strumenti di analoga natura, ad una commissione mista, che opera mediante la redazione di programmi esecutivi pluriennali, a cui è affidata la vigilanza sulla corretta esecuzione degli stessi e l'andamento generale della cooperazione. Questo aspetto è disciplinato, in particolare, all'articolo 15. Il disegno di legge di ratifica consta di quattro articoli. Gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento sono valutati in 33.840 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in 37.740 euro euro annui a decorrere dall'anno 2018 relativamente alle spese di missione, e in 443.500 annui a decorrere dall'anno 2016 per tutte le altre voci di spesa previste. L'analisi della compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con le normative comunitaria ed internazionale cui l'Italia è vincolata. In conclusione, signora Presidente, si propone l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento in esame. **Saluto

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Ne ha facoltà. Signora Presidente, debbo dire che, di fronte ad una relazione compiuta come quella del senatore Lucidi, resta poco da aggiungere. Egli ha ben evidenziato come nei 20 articoli del provvedimento al nostro esame ci sia sostanzialmente una riscrittura di un Accordo precedente. Sottolineo solo che sono passati quasi sei anni dalla firma di questo Accordo e per fortuna ci apprestiamo a ratificarlo in via definita. Desidero ricordare il voto favorevole già espresso dalla Lega alla Camera dei deputati, con l'intervento

Signora Presidente, nel ricordare che la Lega ha già espresso un voto favorevole su questo provvedimento alla Camera dei deputati con un intervento del collega Pini, Credo che sia possibile ribadire anche in questa sede questo orientamento da parte del nostro Gruppo e chiedo l'autorizzazione

scuole dove si insegni l'italiano e di incontri in cui si parli dell'Italia. L'attenzione particolare ai beni culturali archeologici italiani è un fatto che ci fa molto onore. Penso che,

Signora Presidente, come illustrato dal collega Lucidi, il disegno di legge riguarda la cooperazione in materia di cultura e istruzione tra l'Italia e la Repubblica ceca. L'Accordo consentirà di promuovere e incentivare iniziative, scambi e collaborazioni in ambito culturale, scientifico e tecnologico mediante l'organizzazione di convegni e l'attribuzione di borse di studio, facilitando la cooperazione nella conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico e archeologico e e archeologico e inibendo i trasferimenti illeciti di beni culturali. Con questo Accordo favoriamo l'avvio di ricerche congiunte e un'offerta reciproca di borse di studio in settori considerati prioritari. Vengono anche promosse e facilitate le attività delle istituzioni culturali di un Paese all'interno della realtà culturale dell'altro e favorito lo sviluppo di attività comuni tra i propri istituti e le istituzioni culturali del Paese ospitante. L'Accordo disciplina, inoltre, le forme di cooperazione scientifica fra istituti, centri di ricerca e università dei due Stati mediante scambi di documentazione scientifica e tecnologica, scambi di esperienze e di visite di docenti, ricercatori e tecnici. In conclusione, il Movimento 5 Stelle voterà a favore di questo accordo.

all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre Il relatore, senatore Compagna, ha chiesto l'autorizzazione

dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR). Istituita con un accordo sottoscritto nel 1998 da Italia, Francia, Germania e Regno Unito, l'OCCAR è un organismo permanente di gestione comune dei programmi di acquisizione di armamenti. Ai Paesi originari si sono poi aggiunti il Belgio e la Spagna, rispettivamente nel 2003 e nel 2005. Il numero dei Paesi membri dell'Organizzazione è dunque salito a sei, cui devono essere aggiunti altri sei *partner*, la Finlandia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Svezia, la Polonia e la Turchia. Questi ultimi partecipano a singoli programmi dell'Organizzazione, senza tuttavia essere ufficialmente parte della sua struttura istituzionale. Si ricorda che l'articolo 39 della Convenzione riconosce piena personalità giuridica all'Organizzazione, conferendole l'autorità di stipulare contratti, di acquisire e cedere beni mobili ed immobili e di avviare procedimenti legali. L'OCCAR, che ha sede a Bonn, ha il suo organo decisionale nel Consiglio di sorveglianza, composto dai sei Ministri della difesa degli Stati membri o dai loro delegati, che vi partecipano con diritto di voto, ed è presieduto da un presidente eletto dal Consiglio fra i suoi membri. L'organismo decisionale, che si riunisce almeno due volte l'anno, esercita la direzione e il controllo dell'amministrazione esecutiva e di tutti i comitati che il Consiglio stesso istituisce al proprio interno, e decide su tutte le questioni che riguardano l'attuazione della Convenzione. Obiettivo fondamentale dell'OCCAR è quello di coordinare, controllare e realizzare i programmi relativi agli armamenti che le vengono assegnati dagli Stati membri, nonché di coordinare e promuovere attività congiunte

fra cui il Logistic support ship per la realizzazione di una *task force* navale finalizzata a coadiuvare le operazioni di soccorso, a fornire supporto medico e a consentire il trasporto di merci. Le modifiche previste dalla decisione al nostro esame riguardano le procedure decisionali del Consiglio di sorveglianza. La Convenzione prevede infatti in linea generale che tutte le decisioni siano prese dagli Stati membri all'unanimità, fatta eccezione per quelle relative alle materie indicate dall'Allegato IV che sono adottate in alcuni casi a maggioranza qualificata rinforzata, in altri a maggioranza degli aventi diritto. altresì che per quanto concerne le deliberazioni del Consiglio di sorveglianza e dei comitati di programma relative a piani di cooperazione ai quali non aderiscono tutti gli Stati membri dell'organizzazione, la Convenzione prevede che le relative decisioni siano assunte soltanto dai rappresentanti degli Stati partecipanti ai suddetti programmi. L'Allegato IV, al paragrafo l, attualmente prevede che siano assunte a maggioranza qualificata rinforzate le decisioni relative all'ammissione di nuovi Stati membri, alle norme e ai regolamenti dell'OCCAR, all'organizzazione dell'amministrazione esecutiva e alla nomina del suo direttore. Stabilisce inoltre che siano assunte a maggioranza degli aventi diritto di voto le decisioni relative alla istituzione o scioglimento dei comitati. La definizione di maggioranza qualificata rinforzata è contenuta nel paragrafo 1, lettera *a)* dell'Allegato IV, ai sensi del quale «una maggioranza qualificata rinforzata significa che una decisione non può essere presa se vi sono dieci diritti di voto contrari». Attualmente dispongono di dieci diritti di voto solamente gli Stati membri fondatori dell'OCCAR, ossia Italia, Germania, Francia e Regno Unito; a loro volta, il Belgio e la Spagna, membri ma non fondatori, detengono rispettivamente cinque e otto diritti di voto. Il paragrafo 5 dell'Allegato IV stabilisce inoltre che dopo un iniziale periodo triennale, proprio l'*iter* decisionale possa essere riesaminato alla luce di tutti gli elementi rilevanti. La prima modifica proposta dalla decisione al nostro esame, conformemente a quanto previsto dal richiamato paragrafo 5, riguarda alcuni aspetti relativi alle procedure decisionali introducendo un punto al paragrafo 1 dell'Allegato IV, includendo, tra le decisioni prese da tutti gli Stati membri a maggioranza qualificata rinforzata, anche l'assegnazione all'OCCAR di un programma e l'integrazione di programmi di collaborazione in atto tra gli Stati membri. La seconda modifica include nel novero delle decisioni assunte a maggioranza qualificata rinforzata anche la conclusione di qualsiasi accordo o intesa in conformità con gli articoli 37 e 38 della Convenzione, ovvero di quegli articoli che prevedono la possibilità della cooperazione con Stati non membri e con organizzazioni internazionali interessate a partecipare ad alcune attività dell'OCCAR o a uno o più programmi. Le forme di cooperazione sono disciplinate da appositi accordi oggetto di delibera da parte del Consiglio di sorveglianza. La terza modifica amplia il punto che prevede tale maggioranza per la nomina del direttore, richiedendo la maggioranza qualificata rinforzata anche per la nomina del vicedirettore dell'amministrazione esecutiva dell'organizzazione, in considerazione del fatto che in assenza o impedimento del direttore, è proprio il vicedirettore a essere chiamato a sostituirlo. La quarta modifica, infine, signora Presidente, dispone la sostituzione del paragrafo 5 dell'Allegato IV, prevedendo che l'Allegato stesso possa essere rivisto previa decisione unanime del Consiglio di sorveglianza a livello ministeriale. Lo scopo dell'accordo di cui discutiamo è quello di incrementare la cooperazione multinazionale sui programmi di armamento al fine di mantenere e incrementare l'efficienza delle nostre Forze armate in tempi di ristrettezze economiche, favorendo altresì l'adesione alla struttura istituzionale dell'OCCAR di nuovi Stati, soprattutto quelli che già partecipano ai programmi dell'organizzazione. Ovviamente le attività di questo organismo devono essere improntate a criteri di trasparenza, nel pieno rispetto delle norme interne in tema di commercio di armi (per noi, in particolare, la legge n. 185 del 1990). Il disegno di legge di ratifica si compone di tre articoli che riguardano autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore. Non sono previsti costi aggiuntivi o minori oneri. Nella relazione tecnica si evidenzia come l'adesione di nuovi Stati determinerebbe un risparmio sulla partecipazione dei Paesi già membri alle spese di gestione degli uffici dell'organizzazione (che ammontano, per ciascuno Stato membro, a circa 1,7 milioni di euro annui). L'Accordo, signora Presidente, non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e con gli altri obblighi internazionali assunti dal nostro Paese.

perché era uno strumento che garantiva le sinergie migliori e anche il contenimento dei costi in un settore così delicato, ma, ahimè, anche molto costoso per le casse pubbliche. Quindi, è uno strumento che sicuramente va tenuto in adeguata considerazione e le modifiche apportate, in modo particolare il ricorso alla maggioranza qualificata rinforzata in tre casi specifici, vanno nella direzione di rendere ancora più agevole l'adozione di determinate decisioni importanti.

Signora Presidente, vorrei motivare brevemente il nostro voto contrario. Ricordo che all'Accordo istitutivo dell'OCCAR, stipulato tra Italia, Francia, Germania e Regno Unito, hanno aderito successivamente il Belgio e la Spagna, come veniva ricordato, portando a sei il numero dei Paesi membri, ma altri sei Stati, in particolare Finlandia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia, Polonia e Turchia, partecipano a uno o più programmi. Il Consiglio di sorveglianza è il massimo organo decisionale dell'OCCAR e al suo interno sono rappresentanti degli Stati i Ministri della difesa dei Paesi membri che, a loro volta, hanno delegato i rispettivi direttori nazionali degli armamenti.

ha avuto e continuerà ad avere sui meccanismi e sull'efficacia della legge n. 185 del 1990, sull'*export* di armamenti. Voglio ricordare una delle migliori leggi europee nello stabilire il controllo efficace del Parlamento e il divieto di commerciare con Paesi in guerra e che non rispettano i diritti umani. Al contrario, l'accordo istitutivo dell'OCCAR ha trasferito ad un organismo diverso dal Parlamento il controllo sulla gestione dello scambio degli armamenti, con l'aggravante che l'OCCAR ha una personalità giuridica in base alla quale ha assunto completa capacità negoziale: stipula di contratti, assunzione di personale, determinazione di condizioni di attività negoziale in genere. a questo proposito, per quanto riguarda la possibilità di avviare procedimenti legali, la posizione contrattuale dell'OCCAR di cui parlavo sarebbe al riparo di un Accordo internazionale ratificato dai Parlamenti nazionali e quindi in grado di prevalere in sede giudiziaria nei confronti di scelte di livello nazionale, anche dipendenti da ragioni etiche che vadano contro i suoi interessi.

spesso dalla Rete italiana per il disarmo, figurano tra le aziende che approfittano del fiorente mercato e della militarizzazione delle frontiere europee anche per il contrasto all'immigrazione traendo, riteniamo in maniera assolutamente immorale, ulteriori enormi guadagni anche dalle crisi dei rifugiati.

(lo abbiamo visto con l'elezione di Trump), ma ciò che non cambia è l'attitudine dei burocrati europei a creare scatole cinesi, una dentro l'altra; ci chiediamo perché. Secondo noi il motivo è la volontà di aggirare le leggi attraverso accordi diversi tra Stati europei, che non passano nemmeno dal Parlamento europeo e che non hanno alcun controllo, né da parte dei cittadini, né da parte dei parlamenti. L'OCCAR, come sapete, è stata istituita allo scopo di contribuire allo sviluppo e alla gestione dei programmi di armamento intergovernativi e di facilitare i processi di ristrutturazione delle industrie della difesa europee. Fin qui sembrerebbe non esserci nulla di male, ma approfondendo i compiti di questa organizzazione siamo arrivati alla conclusione che tra gli scopi vi è quello di ridurre o aggirare le normative e le procedure nazionali di controllo delle esportazioni. Attualmente la decisione sulla destinazione finale è responsabilità del Paese in cui si realizza l'ultimo assemblaggio dei pezzi da esportare. Questo Accordo ha delle pesanti ricadute sui meccanismi e sull'efficacia della legge n. 185 del 1990 sull'*export* di armamenti di armamenti (una delle migliori leggi al mondo), che stabilisce un controllo efficace del Parlamento e il divieto di commerciare con Paesi in guerra e che non rispettano i diritti umani. Ciò significa che la posizione contrattuale dell'OCCAR sarebbe in grado di prevalere in sede giudiziaria nei confronti di scelte a livello nazionale, anche dipendenti da ragioni etiche, che vadano contro i suoi interessi. L'Accordo non prevede, inoltre, alcun criterio etico stringente nella scelta dei Paesi, organizzazioni e istituzioni con le quali l'OCCAR intende concludere i contratti, cedere e acquisire tecnologia, forniture e strutture militari, se non il riferimento all'ambito del codice di condotta europea sull'esportazione di armi. In conclusione, l'accordo istitutivo dell'OCCAR è uno strumento per aggirare la legge n. 185 del 1990: una legge depotenziata ulteriormente dalla sottrazione dei programmi di coproduzione militare dalla relazione annuale che il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento, a norma dell'articolo 5 della legge n. 185 del 1990. In una fase storica in cui le aziende europee di produzione di armi continuano a fare enormi profitti con la vendita di armi, ad esempio all'Arabia Saudita, che continua a fare stragi di civili in Yemen, abbiamo visto come il nostro Governo ha già aggirato la 185, in un modo al limite della legge. Su questo tema abbiamo già presentato un esposto alla magistratura, ma con l'approvazione di questo scellerato Accordo non avremo più voce in capitolo. Pertanto, dichiaro il voto fermamente contrario del M5S all'atto in esame e invito i colleghi di tutti gli schieramenti a riflettere bene sulla ratifica di un Accordo che toglie ulteriore sovranità a questo Parlamento e ai cittadini.

in gran parte europei e in parte, come nel caso della Turchia, Paesi che sono in situazioni problematiche sia rispetto all'Europa che rispetto alla proprie dinamiche interne. Io sono convinto, e così il mio Gruppo, che, nel momento in cui si firmano degli accordi, si costringono i Paesi a acquisire una una dinamica di consenso rispetto a dei principi, a dei valori comuni, a dei comportamenti condivisi e anche alla condivisione delle modalità di rispetto degli accordi che si fanno. In questo senso, anche per il dibattito che faremo domani sul tema della Turchia, che è un tema molto caldo, noi riteniamo che questo Accordo vada nella direzione di consolidare e di realizzare un accordo più ampio, che va oltre l'Unione europea, e che, in un momento come questo, è un accordo in più che mette insieme i Paesi piuttosto che dividerli. In questo senso, oltre che per il merito dell'accordo, noi voteremo favorevolmente.

il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera, riguarda l'Accordo tra l'Italia e il Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica. Il Tagikistan vanta già con il nostro Paese alcune collaborazioni a livello universitario, che hanno portato allo svolgimento di importanti missioni archeologiche. L'Accordo è finalizzato a promuovere i rispettivi patrimoni culturali attraverso lo scambio di dati ed esperienze tecnico-scientifiche, nonché ad agevolare ulteriormente la collaborazione nel campo della conservazione, della tutela e della valorizzazione del patrimonio artistico ed archeologico, impedendo i trasferimenti illeciti di beni culturali ed assicurando la protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Il testo, che si compone di un preambolo e di 19 articoli, individua innanzitutto la finalità dell'Accordo nell'impegno delle parti a favorire la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, su basi paritarie e di reciprocità, anche nell'ambito dei programmi promossi dalle Regioni italiane e dall'Unione europea, in particolare nei settori dell'arte e della cultura, dei musei, delle biblioteche e degli archivi, dell'istruzione e della cooperazione universitarie, della scienza e del turismo. articoli, da 1 a 6, dedicati all'istruzione universitaria e scolastica, impegnano le parti a sviluppare scambi di esperienze e conoscenze attraverso seminari, scambi di docenti e corsi di perfezionamento. Una particolare attenzione è prevista per la promozione della conoscenza, della diffusione e dell'insegnamento delle rispettive lingue e letterature, nonché per l'assegnazione di borse di studio a favore di studenti e docenti per la frequenza di corsi universitari o per lo svolgimento di periodi di formazione professionale e artigianale. I successivi articoli sono dedicati alle forme di collaborazione fra le parti negli ambiti culturale e artistico, sportivo e giovanile, in quello dei *media* e per il contrasto al traffico illecito di opere d'arte. Per la collaborazione scientifica e tecnologica tra le università, i centri di ricerca e altri soggetti dei due Paesi, si prevede la realizzazione congiunta di studi, progetti, conferenze, e l'organizzazione di visite reciproche e attività scientifiche. Gli organi nazionali coordinatori dell'attuazione dell'Accordo bilaterale sono i due Ministeri per gli affari esteri, mentre ad una commissione mista, destinata a riunirsi alternativamente nelle due capitali, sono affidati l'esame dei progressi della cooperazione culturale e scientifico-tecnologica e l'impegno a concretizzare programmi esecutivi triennali. Di rilievo è l'articolo 13, che impegna le parti a favorire gli scambi di informazione tecnologica e attività congiunte di collaborazione scientifica finalizzate al trasferimento di tecnologie, facendo salvi i diritti afferenti alla proprietà intellettuale. Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di quattro articoli che ineriscono, rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria e all'entrata in vigore del testo. Gli oneri sono valutati complessivamente in circa 172.000 euro annui. L'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con le normative comunitaria ed internazionale cui l'Italia è vincolata. In conclusione, signora Presidente, si propone l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento in esame. Signora Presidente, ringrazio il collega Lucidi per l'ampia relazione, che credo abbia ben chiarito quali sono i contenuti del provvedimento. Alla Camera il nostro Gruppo si è astenuto, ma dopo uno scambio di pareri anche con il collega Divina, che è un profondo conoscitore dell'area, e soprattutto valutando la realtà di Dushanbe e di tutto il Tagikistan, credo sia giusto che l'Assemblea esprima un voto voto favorevole su questo provvedimento, come ribadirò in sede di dichiarazione di voto; lo anticipo in questa sede perché, effettivamente, si tratta di un Accordo che può dare buoni frutti sia ad una parte e che all'altra.

che riguarda la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica. È, quindi, un fatto positivo sia per l'Italia che per il Tagikistan, in particolare per questo Paese, che oggi dimostra una maggiore apertura a livello internazionale, e questo è positivo. Signora Presidente, l'Accordo tratta temi cari al Movimento 5 Stelle, soprattutto nell'ottica di una cooperazione pacifica tra Paesi volta a valorizzare la cultura e lo scambio culturale che, a nostro avviso, può migliorare le relazioni reciproche e avere importanti ricadute nell'ambito della ricerca e, in maniera indiretta, anche nell'ambito del turismo. Per questi motivi

Il relatore, senatore Bianco, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi

il provvedimento in oggetto, licenziato dalla Camera in prima lettura a fine febbraio 2016 e assegnato in sede referente alla 12ª Commissione del Senato in seconda lettura a marzo, raccoglie in una complessa sintesi ben otto progetti di legge depositati alla Camera. Ricordo che altrettanti erano stati a suo tempo i disegni di legge depositati in 12ª Commissione al Senato. Credo sia opportuno ricordare che la proposta della Camera ha correttamente acquisito le linee di indirizzo in materia formulate dalla commissione nazionale di esperti insediata dal Ministro della salute e presieduta dall'allora presidente del consiglio nazionale forense, professor Alpa. Quanto accennato racconta la storia recente, ma che in realtà risale, ancorché su aspetti più limitati, ad atti della XIII legislatura, testimoniando da una parte la necessità di un intervento legislativo su una materia altamente sensibile sul piano civile e sociale, ma diventata ingovernabile, e dall'altra le oggettive difficoltà ad affrontare i molteplici risvolti di un fenomeno (il contenzioso in sanità) che ha inquinato le pratiche professionali di comportamenti opportunistici a scopo difensivo, che grava di costi inappropriati diretti e indiretti i bilanci della sanità pubblica e privata e, non ultimo, che consuma il rapporto fiduciario tra cittadini, professionisti sanitari e istituzioni sanitarie. Il testo licenziato dalla Camera si fa carico di quella necessità, aggravatasi nel tempo, e propone un'incisiva riforma di sistema che, partendo dalla sicurezza delle cure, qualificata come parte costitutiva del diritto alla tutela della salute, ridefinisce la responsabilità civile delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, innova i profili di responsabilità penale e civile degli esercenti le professioni sanitarie, configura una cornice di obblighi per i contraenti e per le imprese di assicurazione idonea a garantire la certezza dei risarcimenti e delle azioni di rivalsa, introduce nuove misure per lo snellimento, la celerità e l'efficacia delle procedure pregiudiziali e giudiziali relative al contenzioso sanitario. Il provvedimento legislativo supera quindi la logica degli interventi settoriali fino ad oggi perseguita, con il fine ultimo di garantire, nella sicurezza delle cure l'appropriatezza delle stesse, nella certezza del diritto, nella trasparenza delle azioni di gestione e nella qualificazione qualificazione delle responsabilità dei vari attori quel clima di serenità e fiducia tra cittadini, professionisti e istituzioni sanitarie indispensabile a reggere le sfide di una tutela della salute universalistica ed equa. Il lavoro della 12ª Commissione, attraverso una fase di ascolto che ha registrato 44 audizioni e la disamina di circa 400 emendamenti, si è sviluppato nel solco delle proposte fortemente innovative già contenute nel testo della Camera e si è concluso con l'inserimento di modifiche che ne perfezionano ed esplicitano alcuni aspetti e contenuti. Non a caso, il provvedimento parte dalla sicurezza delle cure, intesa come sicurezza del paziente e sicurezza degli operatori, sancendo che è parte costitutiva del diritto alla salute. Ricordo che già la legge di stabilità 2016, ai commi 538, 539 e 540, ha anticipato misure finalizzate a potenziare tutte quelle attività di prevenzione e gestione del rischio clinico nelle strutture sanitarie e sociosanitarie, individuando soggetti e procedure di *risk management*. Il provvedimento in esame completa quel contesto operativo, prevedendo un sistema univoco di rilevazione e trasmissione dei dati relativi a rischi ed eventi avversi, sinistri denunciati e risarciti e modalità assicurative per responsabilità civile, da parte delle strutture sanitarie verso i centri regionali, che raccolgono i dati codificati e li trasmettono all'Osservatorio nazionale buone buone pratiche per la sicurezza dei pazienti, presso l'Agenas, anche al fine di promuovere e modulare, nei contesti organizzativi e professionali specifici, attività educative e formative sulla sicurezza. Vorrei sottolineare la grande rilevanza che assume la disponibilità di un sistema univoco, chiaro, essenziale, trasparente e accessibile di questi dati, detto, per ogni attività programmatica, ma anche per stimare gli indici di rischiosità e su questi ottimizzare i premi assicurativi. La trasparenza dei dati relativi al contenzioso, come emersi dalle attività di *risk management*, viene proposta già nel testo della Camera dei deputati sia come uno strumento che avvicina le istituzioni ai cittadini, migliorandone le capacità e le responsabilità di orientarsi sulle scelte, sia come un'opportunità delle stesse organizzazioni di migliorare le proprie *performance*. Va in questa direzione la previsione di un accesso più rapido e facilitato rispetto alla normativa vigente alle documentazioni cliniche (quelle disponibili in sette giorni) laddove si manifestino interessi giuridicamente rilevanti. Il miglioramento della qualità e della sicurezza delle prestazioni sanitarie è strettamente connesso alla produzione, diffusione e assunzione delle buone pratiche clinico-assistenziali basate sulle migliori evidenze disponibili e delle raccomandazioni previste dalle linee guida. Su questo tema sensibile, avente rilevanti riflessi sulla efficacia e costo-efficacia delle prestazioni sanitarie, la Commissione ha sviluppato una approfondita riflessione al fine di bilanciare due principi di rango costituzionale: da una parte, l'esigenza di salvaguardare i principi di universalismo ed equità nella tutela della salute e, dall'altra, l'esigenza di rispettare l'autonomia e la libertà della ricerca tecnico-scientifica pura e traslazionale e dell'esercizio professionale. Questo è un passaggio che, come è facilmente comprensibile, va al di là del diretto riferimento a condotte virtuose che possono sottrarre i professionisti a profili di punibilità penale, peraltro previsti dal testo, offrendo altresì l'occasione per la costruzione - finalmente - di un sistema nazionale di linee guida aperto al contributo di ogni soggetto pubblico o privato, qualificato e individuato in apposito elenco redatto e verificato dal Ministero della salute, ma responsabilmente Il testo proposto dalla Commissione su questa materia si muove nel solco tracciato dal testo della Camera dei deputati, ma, anche su sollecitazione di numerose comunità scientifiche, individua in modo più analitico i requisiti di trasparenza e di qualificazione tecnico-scientifica dei soggetti abilitati a redigere le linee guida e, soprattutto, riprende e riqualifica in questi nuovi il Sistema nazionale linee guida che, sebbene già istituito con un decreto del Ministero della salute nel 2007, ha progressivamente perso nel tempo incisività e autorevolezza nella *governance* della produzione e diffusione di nuovi saperi e competenze. la norma attribuisce all'Istituto superiore di sanità il compito di individuare e rendere pubblici *standard* metodologici di produzione di linee guida, peraltro già adottati dalla comunità scientifica internazionale, rispetto ai quali valutare l'aderenza delle stesse linee guida prima di pubblicarle sul proprio sito istituzionale. Anche questo può e deve costituire una risposta di sistema a quell'analfabetismo scientifico di ritorno, a quel lassismo sul rigore del metodo della ricerca scientifica pura e traslazionale, a quell'oscurantismo e negazionismo scientifici che ogni tanto affiorano e feriscono i pilastri sui quali si sono sviluppate la scienza moderna e la moderna medicina, ma che soprattutto - questo è ciò conta - fanno male alla salute delle persone. La portata riformatrice del provvedimento in esame non poteva non toccare l'ordinamento penale, anche a seguito di una lunga e travagliata riflessione giuridica sulla cosiddetta colpa medica, che ha trovato il suo ultimo punto di caduta legislativa nell'articolo 3 della cosiddetta legge Balduzzi. Tale norma viene abrogata dall'articolo 6, interamente riformulato dalla Commissione giustizia del Senato, introducendo nel codice penale un nuovo articolo, il 590-*sexies*,

Con l'articolo 7 vengono introdotte profonde innovazioni della responsabilità civile in ambito sanitario: la prima riguarda i due diversi regimi di responsabilità in ragione dei soggetti coinvolti dall'azione di risarcimento. Le strutture sanitarie rispondono per inadempimento contrattuale inversione dell'onere della prova e prescrizione a dieci anni) anche per le condotte colpose e dolose degli esercenti le professioni sanitarie di cui a qualunque titolo si avvalgono come prestatori d'opera. Gli esercenti le professioni sanitarie, a qualunque titolo operanti in strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, qualora direttamente chiamati in causa, rispondono del proprio operato per fatto illecito (*ex* articolo 2043 del codice civile, cosiddetta responsabilità extracontrattuale con onere della prova a carico del ricorrente e prescrizione a cinque anni) salvo che - questa è la modifica della Commissione sanità del Senato - abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione contrattuale assunta con il paziente. La seconda innovazione è contenuta nell'articolo 8, ovvero il tentativo obbligatorio di conciliazione che prevede l'obbligo preliminare di colui che esercita un'azione di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria innanzi al giudice civile di proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente; tale richiesta è condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. Il giudice nomina un consulente tecnico d'ufficio con il compito di conciliare la lite nel tempo massimo di sei mesi e con obbligo delle parti coinvolte di partecipare alla procedura, comprese le assicurazioni; qualora la conciliazione non riesca o trascorso il termine dei sei mesi si va in giudizio, anche ricorrendo al rito sommario. Risultano evidenti gli obiettivi delle innovazioni introdotte in ambito civilistico tese a ridurre la pressione delle azioni risarcitorie direttamente rivolte agli esercenti le professioni sanitarie e a favorire la risoluzione della lite in fase pregiudiziale in tempi rapidi e certi o, in mancanza di conciliazione, di acquisire al processo tutti gli atti prodotti. Sull'azione di rivalsa sottolineo come il comma 1 dell'articolo 9 del testo Camera, riproposto in modo integrale dalla Commissione, definisca una norma chiara e centrale nell'impianto della legge e cioè che l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata dagli aventi titolo solo in caso di dolo o colpa La Commissione ha invece innovato il comma 5 dell'articolo 9, anche sulla base di numerose indicazioni raccolte in tal senso, ripristinando, rispetto al testo Camera, la giurisdizione della Corte dei conti per le azioni di responsabilità amministrativa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria per dolo o colpa grave, in caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta nei confronti della struttura pubblica. Questa scelta, peraltro coerente con l'ordinamento generale delle pubbliche amministrazioni in materia di danno erariale, tra le sue opportunità, oltre a quelle note sull'esercizio autonomo dell'azione amministrativa, del potere riduttivo e della non trasmissibilità agli eredi, salvo l'illecito guadagno, contempla anche quella di evitare il paradosso organizzativo che siano le strutture pubbliche a dover avviare le azioni di rivalsa in sede civile, magari legittimamente usando contro i propri professionisti quelle competenze e conoscenze di prevenzione e gestione del rischio non compiutamente acquisibili, nella prevedibile diffidenza dei professionisti a collaborare collaborare in attività che potrebbero essere usate contro se stessi in un giudizio di rivalsa. La normativa interviene altresì da una parte nel quantificare l'ammontare massimo della rivalsa, in caso di colpa grave, dall'altra nel prevedere contestuali misure di carattere disciplinare incidenti per tempo limitato nelle progressioni di carriera. Anche ai fini della rivalsa, il testo prevede, all'articolo 13, misure che obbligano tutti i soggetti destinatari di una azione di risarcimento, che possa coinvolgere la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, di darne a questi tempestiva comunicazione con mezzi idonei. Una riforma di sistema sul contenzioso sanitario non poteva sottrarsi dall'affrontare in modo organico gli obblighi assicurativi, con l'obiettivo di costruire un sistema certo di ristoro del danno, coerente con il nuovo impianto della responsabilità civile. A tal fine, l'articolo 10 ribadisce che le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo in esse operanti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1228 del codice civile. La Commissione ha integrato il testo del comma 1 approvato con la previsione che le suddette strutture devono altresì stipulare polizze assicurative o adottare analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie, qualora questi siano investiti da un'azione di risarcimento promossa ai sensi dell'articolo 2043. In una logica più generale di equilibrio e solvibilità del risarcimento è stata prevista al comma 3 l'obbligatorietà per gli esercenti le professioni sanitarie, passibili di azione amministrativa della Corte dei conti per danno erariale di rivalsa in sede civile, se operanti in strutture private, di stipulare idonee polizze assicurative per colpa grave e dolo. Il quadro di certezze in questo settore è stato ulteriormente potenziato attraverso l'individuazione, mediante decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero della salute,

con indicazioni specifiche relative alla retroattività e all'ultrattività delle garanzie stesse di almeno dieci anni, ai sensi Per le Regioni che adottano altre analoghe misure per la copertura della responsabilità civile, comunemente note come auto-assicurazione, l'obbligo è di dotarsi di un fondo rischi e di gestire i sinistri con accantonamenti per competenza e non per cassa, proteggendo secondo l'ordinamento vigente tali fondi da misure di esecuzione forzata. Infine, l'articolo 14 prevede l'istituzione di un fondo di garanzia, con una norma legislativa totalmente riformulata dalla Commissione nelle modalità costitutive e di funzionamento - c'era infatti un problema tecnico nella formulazione - finanziato con percentuali di premi assicurativi del settore, per coprire gli eventuali risarcimenti sovra-massimali o le condizioni di insolvenza delle imprese assicuratrici.

è risarcito in riferimento a tabelle uniche a livello nazionale, ricordando che tale questione, aperta dal 2007 senza soluzioni, troverebbe finalmente un punto di caduta nel disegno di legge sulla concorrenza e sul mercato, prossimamente in discussione presso dalla Camera dei deputati introduce nell'ambito del contenzioso in sanità una terza modalità di azione per il danneggiato, quella diretta verso le imprese di assicurazione, ma limitatamente a quelle delle strutture sanitarie e sociosanitarie o verso gli esercenti le professioni sanitarie che operano in libera professione, ovvero in ragione di una obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Risulta evidente il fine di incrementare gli strumenti a disposizione del danneggiato per avviare l'azione di risarcimento, scontando così una probabile accelerazione dei tempi del contenzioso e dei costi diretti ed indiretti connessi proprio ai tempi del contenzioso. Il provvedimento riconduce ed armonizza questo nuovo istituto - se volete paragonabile al modello RC auto - alla disciplina generale in termini di prescrizione, di rivalsa e di partecipazione delle parti coinvolte nel giudizio.

Vengono, infatti, rafforzate le procedure di verifica delle competenze e resi trasparenti i possibili conflitti d'interesse rendendo di fatto disponibili al giudice tutti gli albi presenti a livello nazionale (comma 1) e da aggiornare ogni cinque anni (comma 3). Una modifica Una modifica al testo Camera apportata dalla Commissione referente ha di fatto delineato una disciplina speciale per il contenzioso penale e civile avente ad oggetto la responsabilità sanitaria laddove è previsto che l'autorità giudiziaria affidi sempre la consulenza e la perizia a un collegio costituito da un medico specializzato

L'articolo 16 del testo Camera, non interessato da modifiche della Commissione referente, ha, a mio giudizio, almeno una portata straordinaria laddove prevede che i verbali e gli atti conseguenti alla attività di gestione del rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nell'ambito di procedimenti giudiziari. Ricordo che il nostro sistema di responsabilità penale e civile è fondato sul riconoscimento della colpa e, quindi, proteggere la confidenzialità di atti e verbali ha il significato enorme di riconoscere a questi il perseguimento di interessi meritevoli di protezione di protezione (la prevenzione e gestione del rischio) almeno quanto quelli perseguiti dai poteri d'indagine della magistratura nell'accertamento della colpa. Signora Presidente,

Come spero di avervi rappresentato in una sintesi incisiva, si tratta di una riforma efficace, profondamente innovatrice, ma equilibrata nella tutela di tutti i legittimi interessi in campo.

onorevoli senatrici e senatori, il disegno di legge, intitolato «Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario», tratta una tematica di particolare interesse per i cittadini che fruiscono delle strutture e delle prestazioni sanitarie e per l'intero mondo sanitario. L'impegnativa riflessione, anche emendativa, effettuata in *primis* dalla 12a Commissione del Senato, ha contribuito a rendere ancora più efficace, pertinente e lineare il testo approvato dalla Camera

Il titolo proposto è: «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e responsabilità professionale del personale sanitario». D'altra parte, il disegno di legge affronta il tema della tutela dell'assistito, della sicurezza delle cure, della tutela e sicurezza dei professionisti agendo su più aspetti, quali Viene attribuita la funzione di garante per il diritto alla salute al difensore civico regionale o provinciale (articolo 2); vengono istituiti i centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente; viene disposta la predisposizione e pubblicazione sul sito Internet di ogni struttura sanitaria una relazione semestrale consuntiva degli eventi avversi e delle conseguenti iniziative messe in atto, proprio in logica di trasparenza nei confronti dei cittadini e per una loro matura e consapevole scelta; viene istituito l'osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità (articolo 3). altro aspetto riguarda la struttura organizzativa: viene inserito l'obbligo alla trasparenza delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie effettuate dalle strutture pubbliche e private (articolo 4, comma 1); viene statuito l'obbligo della fornitura della documentazione clinica entro trenta giorni dalla richiesta del cittadino comma 2); viene stabilito che debbano essere resi disponibili da ogni struttura mediante pubblicazione sul proprio sito Internet i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio (articolo 4, comma 3). Si indica inoltre che gli esercenti le professioni sanitarie devono attenersi alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni previste dalle linee guida elaborate dalle società scientifiche e tecnico scientifiche iscritte in un apposito elenco istituito e regolamentato dal Ministero della salute (articolo 5). Si definisce che la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata risponde ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile delle condotte dolose e colpose dei professionisti sanitari di cui si avvale, sia che queste siano rese in regime di dipendenza, ossia in regime libero-professionale o di libera professione intramuraria qualora l'evento - esclusa l'imperizia - sia avvenuto nonostante le raccomandazioni previste dalle linee guida ovvero nel rispetto delle buone pratiche clinico assistenziali. Per l'esercente la professione sanitaria viene inserito nel codice penale l'articolo 590-*sexies* (responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). articolo statuisce che «l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave». evidente che è esclusa la colpa grave quando sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge. indica che l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave. Quanto alla parte inerente le assicurazioni, viene definito l'obbligo per le aziende del Servizio sanitario nazionale, le strutture e gli enti privati operanti in regime autonomo o di accreditamento di essere provvisti di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera per danni cagionati dal personale a qualunque titolo titolo operante presso l'azienda, la struttura o l'ente (articolo 10). Viene definito l'obbligo per ciascun esercente la professione sanitaria di provvedere alla stipula, con oneri a proprio carico di un'adeguata polizza assicurativa, a tutela dei cittadini. Infine, per rispondere a danni subiti dal cittadino assistito si attiva sul fronte civile un doppio binario: la responsabilità contrattuale a carico delle strutture sanitarie che, a mio parere, indica una tutela maggiore del cittadino, aggiungendovi anche la prescrizione decennale la responsabilità extracontrattuale a carico di ogni esercente le professioni sanitarie. Sul fronte penale, il testo prevede l'inserimento dell'articolo 590-*ter* nel codice penale che esclude la colpa grave quando l'esercente la professione sanitaria agisce nel rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali

del riorientamento delle organizzazioni sanitarie, del clima lavorativo e curativo assistenziale a vantaggio di assistiti e professionisti. Al di là degli ulteriori, molteplici e complessi aspetti inerenti la componente giuridica e della magistratura, la componente assicurativa e la componente che inerisce le relazioni tra pazienti, tra professionisti e struttura e tra

Si impostano e sperimentano sistemi a rete, si integrano le diverse offerte sanitarie, si propongono nuovi modelli organizzativi, si chiede agli operatori tutti e ai professionisti sanitari in particolare, di adattarsi a questa difficile quotidianità operativa, di essere propositivi e innovatori, di personalizzare il processo diagnostico terapeutico e il processo assistenziale, di garantire personalizzazione e continuità, tutela e sicurezza anche nell'assunto che il professionista sanitario ricopre una posizione di garanzia nei confronti del malato. Questa complessità ha spesso prodotto situazioni clinico-assistenziali difficili, comportamenti che si scontrano con aspettative sempre più elevate in termini di esiti e risultati da parte degli assistiti e dei loro familiari, aumento esponenziale del contenzioso giuridico. Elementi, questi, che hanno dato origine al fenomeno della cosiddetta medicina e assistenza difensiva che produce inappropriatezza nella risposta ai bisogni degli assistiti, oltre che costi aggiuntivi e rallentamenti nei processi di lavoro. Con l'approvazione di questo disegno di legge si potrà cominciare a contenere il fenomeno della medicina difensiva e si comincerà parimenti a costruire serenità lavorativa per i professionisti, a rafforzare il rapporto di fiducia tra i professionisti sanitari tutti (medici, infermieri, ostetriche, tecnici di laboratorio, di radiologia) e gli assistiti tra professionisti sanitari e l'organizzazione in cui operano. Da questo punto di vista sono particolarmente indicativi - e secondo me fondamentali - gli articoli in cui si afferma che la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività (articolo 1, che la sicurezza delle cure si realizza mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche tecnologiche e organizzative (articolo 1, comma 2); che alle attività di prevenzione del rischio clinico messe in atto dalle aziende sanitarie è tenuto a concorrere tutto il personale che vi opera con un impegno e una condivisione di saperi, di responsabilità e di attenzione nei confronti dei cittadini fruitori del nostro sistema salute. Per tutto questo, l'auspicio dell'approvazione del disegno dì legge e di una rapida conclusione dell'*iter* legislativo.

quello di oggi è un provvedimento estremamente importante, che ha suscitato grandi speranze nei professionisti del settore sanitario e che si rivolge non solo a questi ultimi, ma a tutti gli utenti del Servizio sanitario nazionale, come è stato opportunamente evidenziato mediante la modificazione del titolo. Rappresenta, infatti, un contributo fondamentale per l'efficientamento e la sostenibilità del sistema sanitario, mettendo i professionisti in condizione di operare con tranquillità e serenità, e garantendo, quindi, ai pazienti la migliore cura possibile. Il Parlamento ha saputo ascoltare il mondo delle professioni sanitarie nella formazione di un provvedimento atteso da anni, che rappresenta una garanzia per il mondo medico e interviene in maniera positiva sulla limitazione del contenzioso medico-legale, che assorbe ogni anno risorse ingenti e non assicura la soddisfazione del diritto alla salute dei cittadini. Ripercorrendo brevemente alcuni dei punti fondanti dell'articolato, ci convince la norma secondo la quale le Regioni possono affidare al difensore civico la funzione di garante del diritto alla salute, dando la possibilità a ogni soggetto destinatario di prestazioni sanitarie di adire gratuitamente il difensore per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria; in caso di fondatezza della segnalazione, il garante dispone un intervento a tutela del diritto leso, con i poteri e le modalità stabiliti dalla legislazione regionale. In ogni Regione dovrà essere istituito il centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie i dati regionali sui rischi e gli eventi avversi e sulle cause, l'entità, la frequenza e l'onere finanziario del contenzioso e li trasmette all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità. Quest'ultimo soggetto, istituito ai sensi dell'articolo 3, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sarà anche incaricato del monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure e per la formazione e l'aggiornamento del personale e della predisposizione Assume rilievo l'attività di reportistica in un'ottica di trasparenza che obbliga le strutture pubbliche e private a predisporre una relazione semestrale, da pubblicare anche sul proprio sito Internet, sugli eventi avversi verificatisi all'interno

si stabilisce anche che entro sette giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli aventi diritto, la direzione sanitaria della struttura (pubblica o privata) fornisca la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, preferibilmente in formato elettronico. Vengono stabiliti dei parametri di riferimento per le attività dei professionisti sanitari: si tratta delle raccomandazioni indicate dalle linee guida definite ai sensi dell'articolo 5 del provvedimento, integrate nel Sistema nazionale per le linee guida e pubblicate nel sito internet dell'Istituto superiore di sanità. Tali parametri rappresentano anche un fattore fondamentale fondamentale di valutazione, da parte del giudice, di episodi relativi a presunti reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose a causa di imperizia nell'esercizio della professione sanitaria. La normativa vigente, che questo disegno di legge abroga esplicitamente, esclude la responsabilità in esame per i casi di colpa lieve, qualora, nello svolgimento della propria attività, l'esercente la professione sanitaria si sia attenuto a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. La nuova disciplina qui proposta non opera distinzioni generali tra gradi di colpa, escludendo la punibilità per i casi in cui siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida. Si specifica, inoltre, che la forma di responsabilità civile della struttura è di tipo contrattuale (cioè violazione di uno specifico obbligo) e trova applicazione anche con riferimento alle prestazioni sanitarie in regime di libera professione intramuraria, nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica, in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale e attraverso la telemedicina. Si conferma che la responsabilità civile degli esercenti professioni sanitarie, per i danni derivanti dalle condotte dolose o colpose, è di natura extracontrattuale (deriva cioè dalla violazione del generico obbligo di non ledere alcuno senza che prima della violazione sia possibile l'individuazione di una obbligazione). Per la richiesta di risarcimento di danni derivanti da responsabilità sanitaria, la mediazione obbligatoria ai fini della procedibilità della successiva domanda giudiziale viene sostituita con una consulenza tecnica preventiva, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta Inoltre - cosa molto importante - tale provvedimento contiene una norma che limita la possibilità di azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dei propri dipendenti o di responsabilità amministrativa Riguardo all'importo della condanna al risarcimento dei danni in base ai citati procedimenti, si introduce (con esclusione dei casi di dolo) un limite pari al triplo della retribuzione lorda annua. Per quanto riguarda il capitolo relativo all'assicurazione, il provvedimento conferma l'obbligo per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso i prestatori d'opera, a carico delle strutture sanitarie, pubbliche e private. Si specifica, inoltre, che l'obbligo concerne anche le strutture sociosanitarie e le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria o in convenzione con il Servizio sanitario nazionale. Lo stesso articolo 10 prevede l'obbligo, a carico dei professionisti sanitari che svolgano l'attività al di fuori delle strutture suddette, di assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio della medesima attività. Infine, si introduce l'obbligo per gli esercenti attività sanitaria, operante a qualsiasi titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, di stipulare un'adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile per colpa grave. Per concludere, Presidente, mi sembra opportuno ringraziare tutti coloro che hanno contribuito ad un lavoro estremamente complesso, a cominciare dai commissari della 12a Commissione, che hanno iniziato l'esame del testo nello scorso mese di febbraio, conclusosi solo pochi giorni fa in un pacchetto di norme veramente Spero anche che il successivo esame della Camera dei deputati possa avvenire in tempi rapidi, considerando anche che le problematiche regolate dal testo in esame sono strettamente connesse a quelle affrontate dal disegno di legge relativo al settore sanitario, ora all'esame ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

cospicua di disegni di legge di diverse forze politiche. La prima forza politica è stata quella cui è iscritto il mio collega, onorevole Benedetto Fucci, poi se ne sono aggiunte anche altre. In seguito, una apposita commissione ristretta ha provveduto a stendere un testo unificato, nel quale sono confluite le sintesi derivanti da un dibattito che si è appunto svolto in quella sede.

del confronto, dell'approfondimento serio, e non finalizzato a una stucchevole ritualità nelle competenti sedi, prima in Commissione e poi nell'Aula, è un elemento fondamentale. Esso restituisce, non soltanto dignità alla politica, alla politica, ma anche una migliore qualità della produzione legislativa che noi consegniamo al Paese e della quale, purtroppo, troppo spesso, soprattutto in questi ultimi tempi, mi par di capire che ci pentiamo. La misurazione degli effetti della produzione legislativa nel vissuto quotidiano della nostra comunità, infatti, appare sconsolante. Noi abbiamo seguito con attenzione il lavoro svolto alla Camera. Esso è stato orientato a una forma di collaborazione che ha poi prodotto il risultato del testo che noi abbiamo ereditato al Senato e che abbiamo analizzato, valutato, studiato e dibattuto anche con onestà intellettuale. Mi sarei aspettato qualcosa di più, e spero che l'Aula provveda a recuperare quel *quid* che è mancato. Tuttavia, non posso assolutamente ignorare ignorare quanto faticoso sia stato il lavoro del relatore, quanto sia stata brava la presidente De Biasi nel coordinamento dei lavori e quanto difficili siano state l'analisi e la valutazione di un provvedimento che, probabilmente, avremmo meglio affrontato in un lavoro congiunto delle Commissioni sanità

della Commissione. Parlo, naturalmente, di rapporti che non ho mantenuto io e dei quali so molto poco. So, però, che c'è stato un giusto, necessario e forse anche utile (non so fino a quanto, ma lo capiremo) intervento di altri quindi avuto un metodo di lavoro complessivamente positivo.

in capo al cittadino-paziente si sono evoluti nel corso del tempo. Se solo pensiamo che pochi decenni fa la ricetta medica veniva scritta in latino, vediamo quanta quanta strada si è fatta nel restituire in concreto una posizione di centralità al cittadino, che è il destinatario (oggi anche consapevole e protagonista) della prestazione sanitaria che a lui si intende garantire. abbiamo anche tentato di fare qualche passo in avanti e, anche in quella condizione di incertezza, di insicurezza, se non di cronico timore che ha accompagnato l'attività degli operatori della sanità e in particolare quella del medico, è recuperato qualche punto di virtuosismo. Io ritengo che lo sforzo che si è tentato di fare è stato proprio quello di rimettere in una condizione di equilibrio il rapporto tra il medico e il paziente e non vi è dubbio che quando si recupera un buon rapporto tra medico e paziente il risultato è assolutamente positivo nella qualità, nell'efficacia, nell'appropriatezza e nell'adeguatezza della prestazione professionale che si eroga. questo provvedimento pacifica, chiarisce, consegna qualche elemento di certezza in più al medico in ordine al valore e al significato dell'atto medico; non solo fa passi in avanti per un migliore governo del cosiddetto rischio clinico, ma restituisce (ancorché tardivamente) al cittadino una posizione di protagonismo. La possibilità di avere maggiore trasparenza in tutto il percorso terapeutico, dalla presa in carico fino alla conclusione del percorso assistenziale, la possibilità di richiedere e di ottenere e in tempi assolutamente certi

ristabilito in una logica di rispetto delle regole e di chiarezza dei percorsi,

che spesso affrontiamo quando parliamo in generale delle politiche di *welfare* e della nostra sanità. Mi riferisco a quella pagina che passa sotto il titolo di medicina difensiva, di medicina difensiva, che viene considerata come quell'insieme di comportamenti che il medico pone in essere per mettere in protezione sé stesso rispetto al timore che si pongano in essere atteggiamenti talvolta - diciamolo con franchezza - anche di tipo speculativo, al fine di ottenere un beneficio a fronte di una presunta *malpractice* medica. Per carità, esistono anche casi di evidente colpa che meritano di trovare un più efficace e tempestivo riscontro nell'ambito del diritto al risarcimento da parte del cittadino. Forse, però, abbiamo la possibilità, attraverso questo provvedimento, di vedere ridursi

cento dei medici - riferisce l'Agenas - ha ammesso di praticare la medicina difensiva e il 64 per cento la considera uno strumento che ha garantito la diminuzione delle probabilità di errore, ma allo stesso tempo reputa la medicina difensiva un fattore limitante.

positivi abbastanza bassa, anche se deve essere evidenziato che, nel corso degli ultimi dieci anni, il numero degli accoglimenti positivi delle istanze risarcitorie è aumentato.

Questo disegno di legge senz'altro mira alla riconciliazione, alla rifondazione del rapporto tra operatore della sanità e paziente, in particolare tra medico e paziente; paziente; porta ad una sorta di rinascimento della sanità italiana, che ha bisogno di qualcosa in più di un semplice intervento di ammodernamento, e ha

credo siano una pietra miliare, così come la garanzia di terzietà, che si consegue attraverso la previsione del difensore civico, del suo ruolo di garante, dell'apertura

avere contezza di quale sia il contenzioso di una determinata struttura; la possibilità di richiedere l'accesso ai dati di propria pertinenza e di ottenerli in tempi assolutamente ragionevoli. Prima era

che il Ministero adotti un decreto per stabilire i requisiti, ma viene anche palettato il compito del Ministero stesso - e questo mi fa piacere - recuperando ancora una volta l'autonomia che il Parlamento declina attraverso l'approvazione di questo provvedimento. In sostanza, si stabilisce cosa deve contenere il decreto del Ministero: lo *status* giuridico dell'ente o dell'organizzazione che fa le linee guida; la natura giuridica dell'ente; il possesso e il mantenimento dei requisiti e i compiti dell'Istituto superiore di sanità, che ha la

devono essere costantemente aggiornate, recuperando il principio che la medicina non è una scienza esatta, ma è una scienza che si aggiorna con il tempo. Molto spesso la velocità di acquisizione dei prodotti della ricerca scientifica può essere superiore all'aggiornamento delle stesse linee guida; e questo naturalmente viene previsto, disciplinato e codificato.

l'esonero di una responsabilità professionale quando essa è determinata da imperizia e allorquando l'imperizia è accompagnata anche dalla documentata e puntuale testimonianza di aver seguito pedissequamente quanto in ordine al percorso assistenziale quel medico deve osservare in termini di obblighi previsti dalle linee guida. Credo che questo abbia un effetto positivo sotto il profilo deflattivo della quantità cospicua di contenzioso in ambito giudiziario e penale. L'aver recuperato principi più chiari relativi all'azione di rivalsa, con riferimento anche al soggetto che deve avere la responsabilità delle valutazioni (si riporta la competenza al pubblico ministero della Corte dei conti), credo sia un fatto assolutamente importante. Si poteva fare di più? Io dico che si può fare di più. E come si può fare di più? Si può fare di più, signor Sottosegretario, signor relatore, colleghi,

buonsenso, che noi riteniamo possano contribuire a fare un passo in avanti domani in Aula provvederò ad illustrare. Ne cito soltanto due, a titolo esemplificativo. Io mi sono chiesto come mai, dopo appena sei anni dall'introduzione del decreto legislativo n. 28 sulla media conciliazione, si prevede all'articolo 8 la puntuale e precisa esclusione della procedura di media conciliazione dall'attività riguardante il contenzioso che si determina in questa materia. Non mi è stata data una giustificazione. Fonti ministeriali mi hanno detto, in modo documentato, che si ha un effetto assolutamente deflattivo con la media conciliazione, anche se ancora oggi non è sufficientemente utilizzata. E poi c'è un altro aspetto. Io mi chiedo per quale motivo il medico

degli emendamenti che ho presentato e che rimetto alla valutazione del Governo, del relatore e dell'Assemblea.

probabilmente non ci si è resi effettivamente conto della portata normativa di questo fondamentale provvedimento Stiamo parlando dei titoli in base ai quali rispondono il medico e il sanitario nel caso in cui la loro condotta abbia provocato dei danni.

per il paziente danneggiato di agire direttamente nei confronti dell'esercente la professione sanitaria. Questo può sembrare un dato, per certi versi, scontato: chi sbaglia paga; si devono individuare il colpevole,

È ovvio che i parenti, i familiari e lo stesso danneggiato alimentino in cuor proprio la voglia di individuare chi sia il colpevole;

veemente da alcuni rappresentanti degli stessi medici. Si tratta di una preoccupazione che non possiamo dimenticare, non possiamo far finta che non esista e dobbiamo dare delle risposte. Non sappiamo se, effettivamente, il provvedimento in esame possa dare delle risposte. L'analisi di un testo di legge, così come è strutturato, complesso e difficile, non sempre lascia presagire le possibili conseguenze.

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, il testo di legge oggi in discussione si occupa di una materia fondamentale, quale il diritto alla salute

nazionale. Fino ad oggi considerato tra i migliori del mondo occidentale, esso è però messo a rischio per quel che concerne l'universalità, l'equità e la solidarietà, così come si rileva dall'indagine conoscitiva in esame presso la 12a Commissione permanente. Si tratta sicuramente di un problema collegato alla spesa sanitaria, al momento insufficiente ad assicurare l'universalità. Sempre di più, infatti, si assiste al fenomeno dell'abbandono delle cure da parte di una crescente fascia di popolazione. Sempre più assistiamo a una sanità non equa, ovvero non uguale nel territorio nazionale, sempre più si mina il dettato costituzionale sulla uniformità del trattamento sanitario *tout court*. Il disegno di legge oggi in esame contribuisce comunque al miglioramento della sicurezza del nostro Servizio sanitario nazionale. Non c'è dubbio che la sicurezza si realizza con la prevenzione e con la gestione del rischio connesso con l'erogazione delle prestazioni sanitarie e con l'uso appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative. Viene ribadito nel testo di legge che la prevenzione del rischio riguarda tutte le strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, alla quale concorre tutto il personale, comunque e a qualsiasi titolo operante. Si introduce nel disegno di legge la figura del garante per il diritto alla salute, identificandola con il difensore civico, che assume il compito di verificare la fondatezza e la congruità delle segnalazioni provenienti dal paziente o da un proprio delegato. Nello stesso articolo 2, che prevede la presenza del difensore civico, viene prevista l'istituzione del Centro per la gestione del rischio sanitario

in considerazione della composizione della commissione che dovrà elaborarle, porteranno al rispetto dei termini. Bene ha fatto la Commissione sanità a prevedere l'attenersi all'utilizzo delle buone pratiche assistenziali nel periodo di vacanza rispetto all'emanazione delle linee guida e alla pubblicazione delle stesse da parte dell'Istituto superiore di sanità. Novità importanti sono introdotte nell'articolo 6 per quanto concerne la responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria e delle strutture che prevedono l'ottemperamento delle linee guida come parametro di valutazione sull'operato del medico e delle stesse strutture sanitarie. L'introduzione all'articolo 8 del tentativo obbligatorio di conciliazione è un'altra novità prevista nel disegno di legge, che potrebbe snellire il numero delle cause presenti presso i tribunali. Il testo di legge prevede novità sulla stipula di assicurazioni e/o al ricorso di analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi nella forma contrattuale per le strutture sociosanitarie ed extracontrattuale per i professionisti. L'estensione delle garanzie (dieci anni precedenti la conclusione del contratto assicurativo) riteniamo sia operosa per le strutture pubbliche, ma soprattutto per le private, soprattutto di media e piccola dimensione. Auspichiamo, comunque, che questo provvedimento, nel disciplinare i contratti assicurativi, porti a una riduzione dei premi assicurativi che sempre più incidono sui costi delle strutture sanitarie. Particolarmente interessante è la costituzione di un Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, che garantisce il paziente nei casi previsti dalla presente legge per l'insolvenza da parte di società di imprese assicurative e anche per un'eventuale loro messa in liquidazione. Sul risarcimento si introducono sistemi riferiti a un sistema tabellario che rende più equo l'indennizzo.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questo disegno di legge vorrei fosse chiaro che stiamo parlando di disposizioni in materia di responsabilità professionale, ma ritengo anche e soprattutto di disposizioni in materia di sicurezza del paziente. Sono così convinto che questo disegno si debba incentrare soprattutto sulla sicurezza del paziente che proporrò di nuovo, emendamento, il suo inserimento nel titolo dello stesso disegno di legge. In questa discussione generale sono soprattutto due i temi che vorrei affrontare e sui quali mi soffermerò.

andrebbe tenuto presente che le linee guida hanno innanzitutto un valore di orientamento culturale per chi fa medicina. Sono degli strumenti strumenti di aiuto nelle decisioni del medico e non delle regole che devono essere applicate in maniera deterministica. Tale impostazione forse non risponde perfettamente alla visione giuridica delle linee guida della magistratura, ma è coerente con quanto viene sostenuto nel progetto dell'Evidence-based medicine, dove si chiede al clinico di trovare una sintesi tra i risultati della ricerca scientifica e le aspettative valoriali e le peculiarità del paziente che ha di fronte. fronte. Molte volte ci troveremo di fronte pazienti che non hanno una singola patologia su cui poter applicare perfettamente le linee guida. Si tratta spesso di pazienti polipatologici per cui dovremo decidere la linea guida prevalente da seguire. Non esistono delle linee guida che corrispondono a tutte le patologie che in quel momento presenta il paziente. certamente risponde a un sentimento radicato tra i medici, preoccupatissimi molte volte di essere costretti ad aderire a norme vincolanti e a intrusioni esterne nell'autonomia prescrittiva. Pensiamo anche alle dure reazioni che ha suscitato il cosiddetto decreto Lorenzin sull'appropriatezza. Se tra gli obiettivi di Governo e Parlamento c'è anche quello di evitare una grave frattura con i medici, oltre tutto in contrasto con una teoria, dell'accezione internazionale delle linee guida è meglio tenere conto. Dobbiamo partire da un fatto principale: la qualità delle linee guida non è sicuramente garantita dai produttori, non è garantita sicuramente dalle case farmaceutiche e non sarà garantita sicuramente nemmeno dalle società scientifiche. E anche se si tratta di soggetti autorevoli, questa qualità è fondamentalmente legata al rigore metodologico nella fase di elaborazione e, soprattutto, alla *governance* dei conflitti d'interesse che possono influenzare tutto il percorso, dalla formulazione fino alle raccomandazioni cliniche. Dobbiamo altresì tenere presente che all'Istituto superiore di sanità viene assegnato esclusivamente il ruolo di supervisore e di validazione della qualità delle linee guida e della loro trasparenza. Superate queste fasi, le linee guida saranno pubblicate sul sito Internet del Sistema nazionale linee guide (SNLG). Tutto ciò premesso, l'importanza e il potenziale ruolo di indirizzo delle linee guida sono direttamente collegati alla qualità della metodologia seguita nella loro preparazione. E uno dei punti chiave nella loro preparazione risiede proprio nella partecipazione, e anche per questa ragione le agenzie e gli organismi tecnici e indipendenti responsabili di produrre linee guida per il Servizio sanitario nazionale negli altri Paesi coinvolgono gruppi multidisciplinari nel processo di produzione, di designazione e anche di valutazione dei risultati ottenuti. Solitamente includono esponenti degli ordini professionali, degli ordini dei medici, dei farmacisti ed esperti in metodologia con una collaudata esperienza nella produzione delle linee guida; rappresentanti delle società scientifiche e anche delle organizzazioni dei pazienti e i cosiddetti *caregiver*, altre figure eventualmente interessate dal problema oggetto di approfondimento. Quindi, il processo della produzione delle linee guida ha nell'indipendenza dei singoli partecipanti al *panel* degli estensori la principale garanzia di qualità del prodotto finale. E l'indipendenza di questi soggetti da interessi di tipo economico, politico e religioso deve essere garantita da un percorso trasparente e aperto a ogni possibile verifica. A questo punto voglio entrare nel discorso legato alla professionalità e alla responsabilità professionale, che vuole dire molte volte anche elaborare e individuare gli strumenti più idonei sia per valutare quanto fatto, sia per migliorare ciò che si deve fare. Questo provvedimento dovrà incidere a lungo sulla responsabilità della professione sanitaria, sulla sua tutela e sulla sua sostenibilità. Un'organizzazione sanitaria è in grado di garantire cure di qualità in sicurezza solo se implementa un sistema di *risk management*, vale a dire di gestione del rischio. In una logica della prevenzione delle perdite, la cosiddetta *loss prevention*, il *risk management* in un'organizzazione sanitaria rappresenta il nodo fondamentale nella strategia di approccio alla gestione del rischio d'impresa ovvero nell'erogazione di prestazioni sanitarie come una risposta coerente al bisogno di salute, espresso o inespresso, dei cittadini. Questo è il motivo per cui le attività di *risk management* e quelle del comitato di valutazione dei sinistri in un'organizzazione sanitaria devono essere sinergiche. Infatti, se non tutti gli eventi avversi sono sinistri necessitando comunque di un'attenta valutazione al fine di poterne impedire il riaccadimento - è altrettanto vero che non tutte le richieste di risarcimento risultano tecnicamente fondate, anzi la maggior parte di queste è. Le due analisi, però, devono comunque portare ad un miglioramento continuo delle prestazioni. Così come le attività del comitato di valutazione dei sinistri, anche l'approccio del *risk management* deve essere sistemico e sistematico, prevedendo: la fase di *risk management*, ovvero la valutazione del rischio; la fase di *risk evaluation*, e cioè l'evoluzione del rischio; la fase di pianificazione e monitoraggio dei risultati; la fase degli eventuali eventi avversi occorsi e, in questo caso, anche la rivalutazione del processo per identificare eventuali nodi di guasto. È chiaro che le attività del *risk management*, al fine di comprendere il rischio, devono essere progettate con un processo gestionale trasversale e multidisciplinare, che permetta alle organizzazioni di identificare i pericoli correlati ai propri processi produttivi e organizzativi e quantificare la probabilità di accadimento di un evento avverso; progettare le barriere per la contenzione del rischio e di tali eventi e, infine, monitorare i processi e le relative barriere progettate al fine di intercettare situazioni di criticità, implementando così la sicurezza delle prestazioni erogate a garanzia di tutti. In pratica, si pensi all'importanza dell'appropriata gestione del consenso informato, che deve prevedere che che il percorso dell'efficace informazione al cittadino sia non solo trasparente, ma anche ottenibile con la descrizione dei rischi intrinseci ed estrinseci di una prestazione. Per questo credo che la documentazione debba permettere la tracciabilità di tutte le fasi, in termini sia di qualità che di quantità delle informazioni,

Signor Presidente, signor Sottosegretario, relatore, egregi colleghi, il provvedimento in esame è stato approvato alla Camera lo scorso gennaio ed è stato profondamente modificato al Senato nella 12a Commissione per per alcune contraddizioni e illogicità giuridiche, oltre che per alcuni punti su cui potevano esserci dubbi circa profili di incostituzionalità. Tuttavia, ritengo che il testo abbia bisogno di qualche intervento per migliorarne taluni aspetti, e su essi ho ritenuto di presentare alcuni emendamenti. Gli articoli più importanti sono certamente quelli da 5 a 10. La previsione della doppia natura della responsabilità - la responsabilità contrattuale per la struttura ed extra contrattuale per il medico - determinerà inevitabili ripercussioni sulla finanza statale, atteso che con la formulazione attuale della norma le ASL si troveranno a dover sopportare interamente il peso dei sinistri, non potendo ottenere dal medico - o meglio, dalla sua assicurazione - alcun contributo o partecipazione proprio per il diverso titolo di responsabilità per il quale dovranno essere chiamate a risarcire il danno. Sul tema interverrò in seguito con maggiore precisione e dettaglio. Circa il limite al risarcimento dei danni, è stato operato un richiamo alle norme che regolano il risarcimento dei danni da circolazione stradale, benché il presupposto della responsabilità sanitaria sia diverso. Infatti, quel limite ha ragione di esistere per calmierare i premi assicurativi laddove esista per l'assicurazione un obbligo a contrarre (cosa che non c'è in questo provvedimento). Diversamente da quanto accade, quindi, nella responsabilità sanitaria, il cittadino paziente non subisce lesione o decede a seguito di un errore determinato da coloro i quali sono preposti, invece, a garantirne la salute. In ragione di ciò non è dato comprendere perché si dovrebbe limitare il risarcimento, creando una franchigia ad esclusivo favore dei responsabili. Una condizione di procedibilità, quella prevista dall'articolo 8, che non solo, a mio modo di vedere, è in contrasto con alcune riforme della giustizia (tema che approfondirò dopo), creando oltretutto una disparità di trattamento tra coloro (strutture e medici) che operano nel comparto sanitario rispetto a tutte le altre categorie professionali, ma che di fatto potrebbe creare una denegata giustizia per poter agire in giudizio, in quanto le parti lese dovranno sopportare costi elevati solo per esperire una consulenza tecnica preventiva finalizzata alla conciliazione. Parimenti, le strutture sanitarie e i medici coinvolti dovranno accollarsi i costi delle proprie difese legali e tecniche, al fine di tentare di addivenire ad una conciliazione senza avere alcuna certezza che all'esito della consulenza esistano le condizioni economiche per poter affrontare una transazione, mentre la mediazione che esiste oggi costa solo 48 euro, se entro il limite di 250.000 euro, o 80 se supera tale limite, laddove non dovesse riuscire la conciliazione. Penso che questi temi dovrebbero farci riflettere, perché la portata di questo provvedimento probabilmente sta sfuggendo all'attenzione dei colleghi parlamentari, anche perché - parliamoci con grande onestà - il calendario di queste ultime settimane è stato abbastanza leggero. Questo è un provvedimento che ha una portata significativa nei confronti dei pazienti, degli ammalati e dei medici che ha anche implicazioni di carattere giuridico e di carattere economico molto, molto rilevanti. La previsione dell'articolo 8 del disegno di legge complica nuovamente il novero dei riti di procedura civile, appena quattro anni dopo che una riforma era intervenuta semplificandoli, anche nell'ottica della competitività del sistema della giustizia civile. Poi interverrò, signor Sottosegretario e relatore, anche sul tema della deflazione connessa alla conciliazione, perché non sempre i tecnici del Ministero della giustizia riescono ad interpretare i numeri per quello che realmente sono,

il tema della mediazione,

ai colleghi della 12a Commissione e in particolare al Presidente una certa saggezza e equilibrio nel contemperare gli interessi che sono campo e ovviamente voglio auspicare che questi intervengano in una discussione reale e concreta sugli emendamenti che sono stati presentati. Qualcuno sostiene che la mediazione non abbia dato buoni risultati, mi riferisco ai tecnici del Ministero: se questo dovesse essere vero, è certamente conseguenza del fatto che se non fosse stata prevista per legge la partecipazione obbligatoria delle parti probabilmente avremmo avuto risultati peggiori. Sarebbe sufficiente estendere alla mediazione la previsione dell'articolo 8, che prevede l'obbligo di partecipazione alla procedura ivi disciplinata per risolvere a monte la questione, questione, così come sarebbe sufficiente lasciare le parti libere di scegliere se optare per la mediazione o per la consulenza tecnica preventiva di cui all'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile, scelta che può essere certamente dettata dalla consapevole previsione che lo strumento scelto possa essere, nel caso concreto, quello meglio adatto al fine cui è preposta la conciliazione delle parti.

È stato previsto l'obbligo assicurativo per le aziende sanitarie e per i medici, ma non è stato previsto il correlato obbligo a contrarre per le imprese di assicurazione, senza il quale le aziende sanitarie e i medici saranno in balia delle imprese di assicurazione, le quali stabiliranno le tariffe secondo le proprie esigenze e convenienze economiche. Non vorrei, egregi colleghi, che involontariamente si stesse facendo una cortesia alle imprese di assicurazioni.

Ma questa è un'altra storia, a proposito della quale avremo modo di dibattere anche di misure tariffarie e di quale Mezzogiorno intendiamo quando parliamo di diseguaglianze e di sviluppo. Qui, vorrei in particolare soffermarmi, sempre rivolgendomi ai colleghi

sulla vicenda connessa alla responsabilità contrattuale per le aziende sanitarie, pubbliche o private, e alla responsabilità extracontrattuale per l'esercente la professione sanitaria, incluse le prestazioni rese in *intramoenia*, in convenzione e attraverso la telemedicina. telemedicina. Credo che tutti conosciamo quali siano le implicazioni che ciò comporta in termini di prescrizione e di onere della prova. Non vorrei ripeterle, ma quella contrattuale è decennale, quella extracontrattuale è quinquennale. 12a Commissione, dopo un lungo giro di audizioni, ha apportato al testo alcune modifiche prevedendo, in particolare, al comma 3 dell'articolo 7 che l'esercente la professione sanitaria risponde a titolo extracontrattuale, salvo il caso in cui abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale. vorrei fare un piccolo *excursus* sul concetto di obbligazione da risarcimento danni. Il risarcimento dei danni in genere, cioè la norma tipica che disciplina che chiunque cagiona ad altri un danno ingiusto è tenuto a risarcirlo, è quello di cui all'articolo 2043 del codice civile ed è quello classico, che più o meno tutti conoscono, della responsabilità civile da infortunistica stradale. L'elemento che contraddistingue questo genere di obbligazione risarcitoria è che tra chi è che tra chi cagiona il danno e chi lo subisce non vi è, prima del fatto illecito, alcun tipo di rapporto e che l'unica aspettativa o obbligo che esiste tra le future parti del rapporto obbligatorio che va a nascere tra le future parti del rapporto obbligatorio che va a nascere per effetto dell'incidente, è che il primo si aspetta che gli automobilisti rispettino il codice della strada, per fare l'esempio classico del pedone che viene investito o di chi subisce un danno da lesione per incidente automobilistico, e sugli automobilisti grava l'obbligo di rispettarlo e di guidare con prudenza. Questa è la responsabilità extracontrattuale. Quando, invece, tra le parti si stipula un accordo, scritto o verbale, ognuna delle parti assume su di sé un obbligo che, nel caso del prestatore d'opera intellettuale consiste sempre in un servizio che una parte rende ad un'altra in cambio di una controprestazione, in genere somme di denaro. Ho dibattuto a lungo con il relatore, prima ancora che cominciassimo a discutere del provvedimento in Aula, sulla giurisprudenza, di merito e di Cassazione, su quale elaborazione adottare rispetto al tipo di obbligo che grava sul medico e su come sia distinta nettamente l'attività del medico, che è piena di contenuti etici e deontologici, da quella dell'automobilista che ha, invece, il solo generico obbligo di rispettare il codice della strada. Per meglio dire, la giurisprudenza, di merito e di Cassazione, ha distinto il tipo di aspettative che ha il paziente, sapendo che si affida ad un professionista altamente qualificato quale è un medico, da quelle del pedone o di un altro automobilista. Il concetto di affidamento elaborato affidamento elaborato dalla giurisprudenza, sul quale insisto e sul quale ho presentato un emendamento che spero riceva una valutazione attenta, presuppone che il paziente riponga fiducia in chi lo cura, atto cui deve seguire una prestazione qualificata dell'esercente la professione sanitaria che andrà valutata, quindi, *a posteriori*, non con il metro con il quale si valuta il comportamento di un automobilista, ma con quello sicuramente più esigente che si conviene ad un professionista di qualità, nelle mani del quale viene posta la tutela della salute delle persone.

possano sicuramente migliorare alcuni aspetti di questo provvedimento che credo necessitino di maggiore attenzione.

di descrivere in breve lo spaccato che negli ultimi venti e più anni ha caratterizzato il rapporto tra operatori sanitari e utenti, tra medici e pazienti, portando tutto il sistema ad un'estrema radicalizzazione. un rapporto che in passato ha rappresentato l'impalcatura dell'intero sistema sanitario e che con il passare del tempo si è talmente deteriorato da far traballare e scricchiolare pesantemente l'intero sistema sanitario nazionale.

Gli operatori hanno progressivamente portato l'attenzione più sulla patologia che sul paziente, modificando di fatto, proprio in virtù delle note vicissitudini che abbiamo testé rappresentato, cioè questa enorme incrinatura del

che la medicina avesse abiurato al ruolo primario che le competeva e le compete, come la presa in carico del paziente, l'alleviare la sofferenza, insomma tutte quelle attenzioni che hanno caratterizzato e che dovrebbero caratterizzare il rapporto tra il medico e il paziente, determinando

medico forse per l'alto grado di parcellizzazione delle conoscenze, che ha provocato anche un'abbreviazione della visita in quanto tale e, quindi del rapporto intimo tra il medico e il paziente. Si è arrivati quindi al disagio dell'estraneità, all'assenza di empatia tra il medico e il paziente, alla sfiducia crescente, al risentimento fino all'ostilità. Oggi, dunque, il rapporto che si vive è di sospetto, di delusione da parte dell'utenza, e - consentitemi - di frustrazione, di senso di impotenza, di depressione, di negatività e persino di disfattismo da parte degli operatori sanitari, soprattutto da parte dei medici, ognuno con le sue buone ragioni.

quell'essere scevro da pregiudizi decisionali, quella pacatezza e capacità di ascolto che da sempre hanno caratterizzato questa professione senza avere punti clinici di riferimento e percorsi diagnostico-terapeutici ben definiti da linee guida entro le quali muoversi ed interpretare al meglio quell'etica della cura necessaria e indispensabile a garantire fiducia e successo terapeutico compatibili con la sostenibilità del sistema?

consentisse di costruire fiducia e generasse speranza, perché senza queste prerogative essenziali e prodromiche, sarebbe stato prima di tutto l'utente a rischiare la solitudine e poi anche il medico e l'operatore in genere, con il rischio, a brevissimo, che l'intero sistema implodesse inesorabilmente. Stanti queste doverose premesse, diventava ed è diventato convincimento diffuso bisognasse, una volta per tutte, affrontare il problema della responsabilità professionale e risolverlo in modo, diciamo noi, ragionevole, equilibrato e rigoroso, a tutela dell'utenza e della serenità professionale degli operatori tutti, oltre che a salvaguardia dell'intero sistema sanitario nazionale. Come già abbondantemente considerato, sono state avviate discussioni, molte audizioni, sono stati presentati centinaia di emendamenti, sono arrivate molte istanze da più parti. E anche se qualcuno - in modo, secondo il nostro modesto giudizio, molto maldestro - ha reso dichiarazioni pubbliche, dicendo che gli emendamenti sono stati approvati perché vi è stata una riunione alla Camera di una sola parte politica, non ci siamo

conclusione dei lavori. Abbiamo partecipato a questa approvazione con il contributo di tutte le forze politiche presenti in Commissione igiene e sanità del Senato della Repubblica abbiamo portato, secondo noi, a definizione un buon provvedimento. Ed è proprio in funzione di questo lavoro che vogliamo fortemente ringraziare il relatore,

Vogliamo ringraziare anche il sottosegretario De Filippo, perché è stato costantemente presente ai lavori della Commissione. Si tratta di un tema, come dicevamo, che ha visto introdotte molte significative novità, novità, che hanno apportato modifiche sostanziose al testo venuto alla nostra osservazione dalla Camera, modifiche che consideriamo importanti ed estremamente innovative e che, secondo noi, integrano e completano il testo giunto dalla Camera. Il disegno di legge, almeno per gli aspetti che abbiamo ritenuto fondamentali, si incentra soprattutto su un profilo pubblicistico che riguarda le conseguenze penali dell'atto medico,

se gli eventi siano realmente addebitabili non solo al sanitario che viene accusato. È infatti intuitivo che nel campo della responsabilità sia fondamentale l'apporto di periti e CTU, i quali possono illustrare i termini scientifici della fattispecie oggetto del giudizio. È, appunto, sotto questo profilo che ci piace ricordare come il testo apporti modifiche molto importanti, nel senso di un maggiore rigore qualificante nel conferimento degli incarichi.

guida, disciplinate con particolare precisione, sia quanto ai soggetti legittimati ad emetterle, sia con riferimento al loro aggiornamento e alla loro accessibilità.

l'operatore deve considerare sempre le esigenze concrete del paziente, avendo riguardo al fatto che talvolta le linee guida hanno una matrice economico-gestionale e possono porsi in contrasto con alcune peculiari necessità del malato.

l'esercente la professione sanitaria farà in primo luogo ricorso alle linee guida e solo in subordine, in mancanza di raccomandazioni, si atterrà alle buone pratiche clinico-assistenziali. l'osservanza ovvero l'inosservanza delle linee guida non determina né esclude automaticamente la colpa del sanitario. Ciò perché le linee guida rappresentano sì un valido ausilio scientifico per l'operatore, ma non fanno venir meno l'autonomia del professionista nelle scelte terapeutiche. La scienza medica è suscettibile di molteplici influenze - il relatore lo sa molto meglio di noi - e spesso si è chiamati a fare scelte caratterizzate da un elevato tasso di soggettività. Nel corso dell'elaborazione di questo provvedimento, abbiamo pensato che la formulazione forse un po' rigida delle priorità cui sanitario deve attenersi

Bisognerebbe relegare al penale soltanto i casi più gravi, anche se nel testo viene tolta l'illiceità per quanto riguarda l'imperizia, e rimettere al giudizio squisitamente civile, con le cautele assicurative del caso (così come in molti aspetti è stato fatto), i contenziosi relativi alla responsabilità professionale medica. Noi abbiamo lavorato fortemente per migliorare questo provvedimento e siamo fortemente convinti di portare a casa un buon provvedimento.

presenta moltissimi aspetti positivi. Voglio iniziare ringraziando il relatore e tutti i membri della Commissione sanità, ma anche delle altre Commissioni, in particolare della Commissione giustizia, oltre che il Sottosegretario alla salute, per il contributo che hanno dato per arrivare in questo momento ad un provvedimento che giudico di grande

questioni già contenute nella normativa precedente; essa quindi fa fare un salto in avanti rispetto alla disciplina generale del funzionamento del nostro sistema sanitario.

La Camera, alla quale va il nostro ringraziamento, ha prodotto un primo documento che ha sfrondato le cose essenziali e poi ha consentito al Senato, soprattutto alla Commissione sanità, di approfondire alcuni temi che erano stati definiti alla Mi soffermo su alcune questioni. In particolare, tengo a sottolineare come si tratti di un provvedimento che non deve essere interpretato come volto unicamente a tutelare l'esercizio della professione da parte degli operatori della sanità. Questo è un aspetto; ma l'aspetto che mi sta più a cuore è il fatto che esso è volto a tutelare il diritto dei cittadini a ricevere le prestazioni sanitarie in caso di bisogno,

con riguardo a questo provvedimento, ma anche in termini generali, persino con riferimento ad eventuali disfunzioni che l'organizzazione dei servizi sanitari può comportare nei confronti di un cittadino che ha bisogno di essere preso in carico. Sappiamo infatti come il monitoraggio dei livelli di assistenza (che è altra cosa, ma che dovrebbe essere uno dei tanti strumenti che ci consente di consente di osservare come i diritti dei cittadini vengono rispettati) sia da riqualificare. Da molto tempo la normativa prevede che il sistema di monitoraggio possa essere riqualificato, inserendo molti indicatori che attualmente non ci sono e aspettiamo

Questa è un'altra questione importante, perché ciò di cui ci stiamo occupando è il rischio legato all'esercizio delle professioni sanitarie e il rischio di eventi avversi. In un mondo che conosce bene tutti i rischi che si corrono in un settore così complesso come quello sanitario, alcune aziende sanitarie e Regioni hanno già iniziato ad avviare centri

debba osservare non soltanto i casi di denuncia, ma anche gli eventi avversi che si verificano e, soprattutto, debba produrre le linee di indirizzo per la prevenzione e la gestione del rischio

ha in sé, le qualificazioni necessarie per svolgere questo ruolo. Si richiama la procedura che è stata inizialmente definita nel 1996 con la legge n. 662 e via via modificata e implementata. Purtroppo, questa procedura è stata seguita molto poco e, soprattutto negli anni più recenti, è rimasta un po' dormiente. Produrre le linee guida - lo sappiamo, è già stato detto - non è così facile e, quindi, bisogna costruire la forza, la reputazione, l'autorevolezza e l'indipendenza di tutti coloro che collaboreranno a questa attività. Desidero sottolineare un aspetto: il fatto che le linee guida vengano prodotte ed elaborate anche dalle amministrazioni pubbliche (da tutte le amministrazioni ed enti di ricerca e non soltanto dalle società scientifiche) è un passo fondamentale che è stato compiuto con il nuovo testo del provvedimento. Le società scientifiche possono avere un compito importantissimo, ma sappiamo che il rischio di distorsioni legate a eventuali conflitti di interesse non è dietro la porta, ma proprio davanti.

siano prodotte, promosse e coordinate da un'autorità pubblica, che mi auguro che sia proprio l'Istituto superiore di sanità, in base alle migliori evidenze scientifiche e con la consapevolezza che, una volta definite, dovranno

che le linee guida non saranno prodotte rapidamente; per fortuna, sono indicate anche le buone prassi e si dice anche che le eccezioni sono le specificità del caso concreto, quindi non c'è alcun e alcuna perdita di autonomia del professionista, il quale si attiene alle linee guida, importanti per garantire appropriatezza, ma poi deve sempre ragionare in scienza e coscienza. Vorrei

di sfruttare tutte le posizioni dominanti che ha sul mercato, ma non possiamo certo prevedere soluzioni diverse. Dobbiamo essere capaci di conferire alla pubblica amministrazione, alle aziende sanitarie e alle Regioni la forza per negoziare contratti e

sappiamo benissimo che, se questa norma verrà attuata in modo puntuale, potrà recare, nel tempo, beneficio al sistema sanitario, perché ci libererà di tutto quel sovraconsumo di prestazioni che molto spesso viene proposto semplicemente per i timori propri della medicina difensiva, ma sappiamo anche che nel breve periodo, per uno o due anni, questi risparmi non ci saranno, ma ci saranno maggiori oneri. Purtroppo sappiamo che a questo provvedimento non abbiamo potuto affiancare alcun finanziamento specifico. Ci auguriamo che la legge di bilancio, che ha già garantito un aumento di due miliardi di euro per il sistema sanitario, mantenga questo maggiore finanziamento fino alla fine del suo percorso parlamentare, che su questo non ci siano *spending review* e che, quindi, le aziende che si troveranno a sostenere sin da subito maggiori oneri non debbano essere ulteriormente afflitte da restrizioni che, invece, in prospettiva possono migliorare il funzionamento del sistema.

Signor Presidente, nel *weekend* in rete sono state pubblicate le ordinanze di misura cautelare scaturite dall'indagine Amalgama delle procure di Roma e di Genova

Inoltre, tutti ricordiamo le intercettazioni precedenti, in cui il prefetto, sempre di Alessandria, per le questioni legate alle norme antimafia sul Terzo valico, telefonava ad Incalza al Ministero delle infrastrutture e Questi fatti sono gravissimi. Il ministro Alfano deve tutelare la buona immagine degli uffici territoriali del Governo e svolgere tutti quegli atti volti a far sì che le prefetture siano un esempio di legalità e specchiata onorabilità. Ecco perché è necessario che proceda con l'immediata sospensione del vice prefetto di Alessandria e l'immediato trasferimento ad altra sede del prefetto Tafuri. Dalle indagini emergono inquietanti particolari circa l'esecuzione delle opere di questa infrastruttura: si parla di cemento simile ad acqua, simile a colla, eccetera. Giungono, tra l'altro, notizie di alcuni problemi nelle gallerie come in quella di Pontedecimo, a Genova, dove pare che si stia centinando la volta in fretta e furia

quindi a gran voce una immediata sospensione dei lavori nei cantieri incriminati dall'ultima ondata di arresti e l'istituzione di una commissione tecnica che controlli centimetro per centimetro ogni manufatto, ogni gettata di cemento, alla ricerca di eventuali anomalie. Bisogna compiere le opportune verifiche e non andare avanti come un treno - che probabilmente da lì non passerà mai - ad ogni costo. Sarebbe troppo facile, dopo, piangere quando ci saranno i morti. Annuncio che mi accingo a presentare due interrogazioni, una al Ministero dell'interno e una al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per avere risposte su questi argomenti e sollecitare i Ministri competenti perché si attivino immediatamente per porre fine a questa inaccettabile situazione.

con questo intervento di fine seduta continuiamo, oggi, al Senato, una staffetta con cui, assieme a tante senatrici e tanti senatori, ricordiamo ogni donna che viene uccisa per mano di un uomo a cui è o è stata legata da relazione amorosa. Lo faremo sino a quando sarà necessario ricordare al Parlamento e al nostro Paese l'urgenza di arginare la violenza nei confronti delle donne: qualsiasi tipo di violenza, fino a quella più drammaticamente estrema, che comporta la privazione della vita. Non possiamo e non vogliamo abituarci a questo. A Sassari una donna, Anna Doppiu, di sessantaquattro anni, è stata selvaggiamente picchiata dal marito, che poi l'ha bruciata ancora viva. Non se l'era sentita di denunciare il marito, da cui subiva violenze e dal quale, peraltro, aveva deciso di separarsi.

investita dal *camion* guidato dall'uomo con cui aveva questa relazione. L'uomo adesso è in stato di arresto, con l'accusa di omicidio volontario. Salgono così a 26 le donne che abbiamo ricordato in questa staffetta, iniziata solo il 30 giugno. Sono tante le persone che a Sassari, lo scorso sabato, hanno partecipato ad un *flash mob* in cui sono state ricordate, oltre ad Anna, le 98 donne vittime di femminicidio nel solo 2016, così come sono tantissime le persone che a Siena, in questi giorni, hanno partecipato alla fiaccolata in ricordo di Ionela. L'ISTAT ci informa che In Italia ogni 2,2 giorni viene uccisa una donna. Il 46,3 per cento delle donne uccise muore per mano del suo compagno. Il drammatico bollettino risulta ancor più grave per il fatto che le violenze fisiche e sessuali sono ulteriormente aumentate e che sono in crescita anche i casi di violenza assistita. Come dimostrano anche i casi di Anna e di Ionela, il femminicidio è quasi sempre l'estremo risultato di una serie di comportamenti violenti di lunga data. Non serve solo l'attenzione e la consapevolezza di essere di fronte ad un problema da affrontare con decisione, ma è necessario dare tutela, sostegno, risposte e aiuti concreti a tutte le donne che vivono situazioni di potenziale pericolo. Bisogna agire con severità e con un monitoraggio costante di tutte le situazioni a rischio, per non lasciarle incancrenire. Donne e uomini insieme possono fermare questa carneficina. Lo possono fare chiedendo l'applicazione rigorosa delle normative, ma avendo anche la forza di innescare quel cambio di passo, *in primis* culturale, che consenta di sostenere e far vivere la parità di genere dappertutto, in ogni settore, di promuovere l'educazione dei figli, nell'ambito scolastico e famigliare, al rispetto del corpo delle donne, unitamente al fatto che figlie e giovani donne devono trovare la forza di avere più rispetto per sé e per il loro corpo, denunciando la violenza fin dalle prime quasi impercettibili mosse, senza mai giustificarla. La società e le istituzioni debbono essere in grado di rispondere subito alla minima richiesta di aiuto e di assistenza. Abbiamo bisogno di una democrazia paritaria e che affermi i diritti, per scardinare una cultura che è ancora patriarcale, per fare prevenzione, per sconfiggere stereotipi sessuali e pregiudizi, per garantire le libertà e l'autonomia di scelta nel percorso di vita delle donne. Riproponiamo con convinzione il nostro appello. Un appello alla Ministra per le pari opportunità e al Governo tutto: la cabina di regia verifichi costantemente l'applicazione, i pregi e i limiti della legge n. 119 del 2013 e, soprattutto, dia piena e accurata attuazione del piano contro la violenza. Un appello ai *media*: si smetta di giustificare gli assassini e di colpevolizzare le donne. Un appello al Paese, uomini e donne:

voglio tornare indietro nel tempo di una settimana circa e rivivere con voi l'elezione di Donald Trump a Presidente degli Stati Uniti d'America, intanto, per rivolgergli i migliori auguri di buon lavoro a nome degli italiani residenti negli USA e, poi, per focalizzare l'attenzione su un dato in particolare. Anche in Italia, così come negli Stati Uniti, l'elezione di Trump è stata accolta con troppo stupore dalla stampa più influente.

sulla vittoria di Hillary Clinton, un po' come hanno fatto le principali emittenti americane nell'ultimo mese di campagna elettorale, seppur con un tono leggermente più prudente rispetto a quanto letto e visto in Italia. Gli organi di informazione non dovrebbero neppure pensare ai sondaggi. Dovrebbero invece informare, spiegare realmente come stanno le cose, anziché provare a influenzare il voto e l'opinione pubblica. Da cittadino americano ho vissuto in prima persona le elezioni presidenziali dello scorso 8 novembre e, ancora una volta, sono stato fiero di aver contribuito con il mio voto all'esercizio della democrazia, perché il voto della gente, del popolo è un diritto ed è sempre frutto della democrazia. Per le strade delle principali città americane il termometro politico segnava temperature diverse da quelle registrate da sondaggisti e opinionisti, troppo impegnati a inseguire l'*audience* anziché ascoltare la gente. Il voto, invece, non perdona; non è frutto di supposizioni, ma è la concretizzazione di un'ideale, di una protesta o della semplice voglia di cambiare. cambiare. Quando si pensa troppo alla politica e ci si illude che occupare spazi televisivi e pagine di giornale possa radicalmente cambiare le convinzioni delle persone, spesso si va a sbattere contro il muro della sconfitta. Noi che facciamo politica e che rappresentiamo il popolo abbiamo il dovere di informare e di ascoltare chi ci vota. Prima di provare a cambiare il Paese, dovremmo capire in che modo la nostra gente vorrebbe il Paese del futuro. Ricordiamocelo bene, perché tra pochi giorni tutti noi parteciperemo a un altro grande e straordinario esercizio di democrazia: il *referendum* costituzionale. I sondaggi dicono tanto e niente. Le risposte le daranno gli elettori e speriamo di aver compreso bene le loro richieste e il loro pensiero.